Onorevole Presidente, Le trasmetto il messaggio con il quale chiedo alle Camere una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, in ordine alla legge: "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo", approvata dal Senato della Repubblica il 6 ottobre 2016 e dalla Camera dei Deputati il 3 ottobre 2017. Voglia gradire, Onorevole Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. *f.to* Sergio Mattarella». Do quindi lettura del messaggio inviato alle Camere dal Presidente della Repubblica: Onorevoli Parlamentari, mi è stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo". Il provvedimento (che si compone di sette articoli) è stato approvato dalla 6a Commissione permanente del Senato in sede deliberante il 6 ottobre 2016 e, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2017. Con esso, si introduce, all'articolo 1, per gli intermediari abilitati (come definiti dall'articolo 2), il divieto totale al finanziamento di società, le quali, in Italia o all'estero, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgano attività in qualsiasi modo connesse alla produzione ovvero alla distribuzione o commercializzazione di mine antipersona, munizioni e submunizioni *cluster*. La legge contiene aspetti innovativi, che risultano indubbiamente positivi giacché potenziano le misure di contrasto alla produzione di tali pericolosi e insidiosi ordigni bellici, prevedendo, tra l'altro, la responsabilità amministrativa a carico degli enti. Al contempo, deve rilevarsi la presenza al suo interno di una disposizione che risulta in evidente contraddizione con le dichiarate finalità dell'intervento normativo e che appare connotata da rilevanti profili di criticità. Mi riferisco all'articolo 6, rubricato "sanzioni", che al comma 2 priva di rilevanza penale le operazioni di finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti che rivestono posizioni apicali all'intero degli enti intermediari abilitati. In tale comma, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. La materia oggetto della citata disposizione è già regolata, in via generale, da norme penali contenute nella legge n. 374 del 1997 e nella legge n. 95 del 2011. Quest'ultima prevede la messa al bando delle *munizioni a grappolo* e ratifica e dà esecuzione alla Convenzione di Oslo (fatta a Dublino il 30 maggio 2008), incriminando all'articolo 7 l'assistenza finanziaria in favore di chiunque impiega, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse e sanzionando tali comportamenti con la reclusione da tre a dodici anni e la multa da euro 258.228 a euro 516.456. La condotta di "assistenza finanziaria" (contemplata tra quelle vietate dall'articolo 1 della Convenzione di Oslo) è quindi perfettamente sovrapponibile a quella proibita dall'articolo 1 della legge in esame, per la quale viene prevista soltanto la sanzione amministrativa dall'articolo 6, comma 2, se realizzata dai soggetti qualificati sopra indicati. Per ciò che riguarda le *mine antipersona*, l'articolo 7 della legge n. 374 del 1997 sanziona, con le medesime pene, chiunque usa, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene le stesse mine antipersona o parti di esse, ovvero ne utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero. Tale disciplina è espressamente fatta salva dall'articolo 9 della legge n. 106 del 1999, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 1997. Il finanziamento concesso per le attività vietate dal suddetto articolo 7 integra uno dei comportamenti contemplati dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Ottawa, che impegna in modo esplicito gli Stati a vietare, tra l'altro, di "assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque ad intraprendere" le attività proibite dalla stessa Convenzione. Le due previsioni incriminatrici sono il frutto dell'attuazione di obblighi internazionali contenuti nelle Convenzioni, ratificate dall'Italia, le quali esplicitamente richiedono, entrambe all'art. 9, l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse. Pertanto, il loro nucleo normativo non può venire modificato senza che ne risulti leso direttamente il principio tutelato dall'articolo 117 della Costituzione, il quale prevede l'obbligo di esercitare la potestà legislativa "nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". La Corte Costituzionale sin dalle sentenze numeri 348 e 349 del 2007 ha chiarito che l'articolo 117 della Costituzione è idoneo ad attribuire una posizione particolare nel sistema delle fonti alle norme internazionali quali norme interposte in un eventuale giudizio di costituzionalità, sicché le leggi che contrastino con Trattati internazionali che hanno già avuto esecuzione nell'ordinamento interno sono viziate per incostituzionalità. Da ciò deriva una forza delle leggi di esecuzione dei menzionati Trattati tale da escludere che le condotte di assistenza finanziaria alle attività proibite possano rimanere prive di sanzione penale e ciò al fine di assicurare che la violazione del divieto sia efficacemente contrastata. Sul descritto quadro normativo interviene la disciplina contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge in esame il quale non contempla la "clausola di salvaguardia penale" (*salvo che il fatto costituisca reato*). Ciò produrrebbe, in virtù del principio di specialità dell'illecito amministrativo dettato dall'articolo 9 della legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento, poste in essere dai soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionate solo in via amministrativa, in contrasto con gli obblighi internazionali. Tale effetto riguarderebbe non soltanto le future condotte di violazione del divieto di finanziamento, ma anche quelle commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, rispetto alle quali, mancando una disciplina transitoria, non sarebbero applicabili neppure gli illeciti amministrativi (Cassazione penale, Sotto diverso, ma connesso aspetto, debbo ancora segnalare che il venir in essere, per la medesima condotta di finanziamento, di due regimi punitivi diversi - l'uno penale, l'altro amministrativo in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non imprenditore individuale), pone profili di dubbia compatibilità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione. Infatti, le persone fisiche che esercitano funzioni di amministrazione e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, beneficerebbero, per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 6 comma 2, di un regime sanzionatorio solo amministrativo. Viceversa, tutti gli altri soggetti che prestino assistenza finanziaria al di fuori del circuito degli intermediari abilitati (quindi in ragione dell'assenza di un atto amministrativo di autorizzazione) resterebbero soggetti alle sanzioni penali sopra illustrate. Per i motivi innanzi esposti, l'articolo 6, comma 2, del provvedimento presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale. Questi possono essere superati soltanto attraverso un intervento limitato, ma necessario, che assicuri la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, alle attività proibite dall'articolo 1; rilevanza che, per converso, verrebbe irrimediabilmente meno con l'entrata in vigore della legge. Pertanto, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione una nuova deliberazione in ordine alla legge approvata il 3 ottobre 2017. *f.to* Sergio Mattarella *controfirmato* Paolo Gentiloni». Detto messaggio (*Doc*. I, n. 2) sarà stampato, distribuito e trasmesso alle Commissioni competenti. Il disegno di legge n. 57-*bis*, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del Regolamento, dovrà iniziare il proprio *iter* in Senato. In data 26 ottobre 2017, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha inviato la seguente lettera: «ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme

ha eletto in data odierna il dottor Giovanni Amoroso, Giudice della Corte Costituzionale, in sostituzione del dottor Alessandro Criscuolo che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il giorno 11 novembre 2017 per scadenza del periodo di nomina. una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio». Comunico che è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2960, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020». Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di stabilità appare appare nel complesso in linea con le prescrizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, con riguardo al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per le seguenti disposizioni: l'articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale si prevedono modifiche al codice di procedura civile; l'articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza; l'articolo 89, comma 11, che modifica il codice del processo amministrativo; l'articolo 99, relativo all'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo dei rapporti professionali regolati da convenzioni; l'articolo 102, che modifica la tabella recante l'elenco delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dello Stato, al fine di inserirvi l'Associazione nazionale partigiani cristiani. Dispongo pertanto lo stralcio di tali disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge. Deferisco il disegno di legge n. 2960 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) alla 5ª Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni sono pertanto autorizzate a convocarsi o ad integrare i propri ordini del giorno.

ha esaminato gli episodi accaduti nelle sedute di Assemblea del 24 e 25 ottobre 2017. Il Consiglio di Presidenza ha irrogato, con effetto immediato, le seguenti sanzioni, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento del Senato: nei confronti del senatore Santangelo l'interdizione a partecipare ai lavori dell'Assemblea per due giorni *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*; nei confronti delle senatrici Moronese e Taverna la censura e l'interdizione a partecipare ai lavori dell'Assemblea per un giorno; nei confronti dei senatori Airola, Cioffi, Crimi, De Petris, Donno, Giarrusso e Lucidi l'interdizione a partecipare ai lavori dell'Assemblea per un giorno; nei confronti dei senatori Cotti, Ichino, Paglini, Petraglia, Puglia, Russo e Serra la sanzione della censura. Ai sensi del comma 5

Signor Presidente, mi permetto di rivolgere un appello al Governo e ai Capigruppo di maggioranza e chiedo a lei

siano messi nelle condizioni di espletare la propria attività sia la Camera dei deputati che il Senato. Noi abbiamo qui il provvedimento

oggi ha dimostrato senso di responsabilità contribuendo a garantire il numero legale proprio per non ritardare i lavori del Parlamento. Ci auguriamo di riscontrare senso di responsabilità e rispetto

brevemente per lasciare traccia di un'interrogazione che ho presentato al signor Ministro della giustizia in difesa di un imprenditore siciliano, Maurizio Ciaculli, che ha denunciato la presa della mafia sul grande mercato alimentare di Vittoria e che per questo è stato più volte minacciato verbalmente, ma anche materialmente, in ultimo con una lettera anonima contenente minacce di morte e con un sabotaggio della sua vettura. Ciaculli nel 2012 è stato fatto fallire perché una banca locale ha stornato in modo illecito 215.000 euro dalla società che egli dirigeva,

Il punto è che la mafia non è scomparsa. Oggi, signor Presidente, una conduttrice televisiva, Myrta Merlino, si è chiesta come mai parlino così poco di mafia le grandi coalizioni che concorrono

del lavoro toccasse ai magistrati e alle Forze dell'ordine e, con il grosso del lavoro, anche il grosso del rischio, che ha portato alla scia di sangue che tutti conosciamo. Difendere Ciaculli - questo chiedo al Ministro della giustizia - è un modo di dire che non dimentichiamo chi denuncia anche nei posti come Vittoria, dove a denunciare sono molto pochi.

Sono stati esposti dei manifesti, che sono stati anche riprodotti in volantini consegnati casa per casa, da parte della Lega, in cui si mette in relazione il mancato voto al *referendum* del 22 ottobre della sindaca di Casier una relazione che noi sappiamo non esistere - con il fatto di essere impedita, a questo punto, a chiedere alla Regione di fare ciò che deve, e cioè realizzare una infrastruttura che è doverosa ed è stata promessa ai suoi cittadini. C'è però di peggio, caro Presidente: questa sindaca ha visto anche l'esposizione del proprio certificato elettorale, quello che i cittadini del Veneto che sono andati a votare il 22 ottobre hanno ricevuto nei seggi.

tra coloro che hanno scelto liberamente di rappresentare con un non voto la loro posizione e coloro che invece hanno scelto di accondiscendere alla volontà della Lega recandosi a votare. Questo è uno stile che noi conosciamo e che purtroppo si aggrava di giorno in giorno con elementi sempre più rilevanti. La sindaca in questione è evidentemente oggetto, oggi, di una lista di proscrizione,

anche nei confronti degli amministratori pubblici locali. Chiediamo quindi l'intervento del ministro Minniti, affinché proceda a verificare se esistano gli estremi per promuovere azioni nei confronti di coloro che si

Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che sta per iniziare la sessione di bilancio, sarebbe bene che le pubbliche amministrazioni non sperperassero i denari del contribuente. Questo è ciò che accade, invece, al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il cui direttore è stato già condannato a pagare le spese per giudizi inutili, seguiti a suoi illegittimi dinieghi di accesso agli atti. Il direttore ha già perso 2.500 euro per iattanza, arroganza e abuso di potere. Lo dimostra, da ultimo, la sentenza del TAR del Lazio del 30 ottobre 2017, relativa al professor Verrecchia, che aveva domandato l'accesso agli atti

patrimonio dell'UNESCO straordinario, che purtroppo - come è accaduto anche in Piemonte e in molte altre realtà del Nord - in queste ore sono stati oggetto di attentati incendiari.